con lettera del 19 ottobre 2023, il senatore Enrico Borghi ha comunicato che l'Assemblea del Gruppo da lui presieduto ha deliberato la variazione della denominazione del Gruppo stesso in «Italia Viva-Il Centro-Renew Europe». Con lettera pervenuta in pari data, i senatori Gelmini, Calenda, Versace e Lombardo hanno contestato la legittimità della predetta deliberazione. La Presidenza ha pertanto avviato le verifiche conseguenti.

del Governo, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo oggi ad esaminare in Aula è un disegno di legge di iniziativa del Governo, l'Atto Senato 674: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali». un disegno di legge del Governo molto importante in termini non solo di semplificazione, ma anche di regolazione del mercato dei capitali, che ultimamente è un po' asfittico nel nostro Paese. Quindi, il Governo si è posto oggi l'obiettivo di

dell'educazione finanziaria. Si tratta di una norma importante che il Governo ha recepito da disegni di legge che, anche nelle passate legislature, sono stati presentati da numerosi colleghi, che voglio

da coprire rispetto agli altri Paesi europei, in un momento di evoluzione non soltanto del sistema economico e finanziario, ma anche degli strumenti che abbiamo a disposizione. Oggi vediamo che nelle nostre città - e questo è anche un problema - sono sempre meno

motivazioni personali. Mi preme sottolineare insieme alcuni aspetti, anche per chi ci segue. Leggevo oggi, nel venire in Aula,

forza. L'obiettivo fondante del provvedimento in esame, che in sostanza semplifica la possibilità delle nostre imprese di quotarsi sui mercati finanziari, è di mettere in parallelo l'attività dei mercati finanziari con quella delle banche.

sono circa 190 miliardi di euro - nel mentre stiamo mettendo in campo una legge di bilancio che ha pochi spazi di manovra, pari a circa 28-30 miliardi di euro di euro - le risorse degli italiani che direttamente o indirettamente vanno nel capitale di rischio di imprese oltre confine. È questa l'importanza del provvedimento in esame, se proprio vogliamo sottolineare tutti gli aspetti a cui europea ci spinge, con le direttive e anche con l'idea di costruire un mercato dei capitali finanziari europeo, dove si compete complessivamente.

in un momento in cui si parla spesso di Governi che schiacciano la funzione del Parlamento, che la nostra Commissione, in seno a questo Parlamento, ha avuto un grande vantaggio nel confronto con i diversi *stakeholder* che abbiamo ascoltato e le associazioni di categoria, attraverso un emendamento che io e il mio collega abbiamo voluto presentare per smuovere l'aspetto più controverso di questo provvedimento: mi riferisco alla garanzia delle minoranze nei consigli di amministrazione. Sulla base di tale emendamento il Governo, che ha lasciato campo libero al Parlamento per intervenire, ha avuto un testo di riferimento con cui minoranze e la maggioranza, con le sue diverse sensibilità, hanno messo in campo un testo che credo rappresenti la misura di equilibrio migliore possibile che ha accompagnato il dibattito.

davvero il Governo, tramite il sottosegretario Freni, per la libertà con cui tutto il Parlamento, anche la minoranza, si è espresso nell'emendare al meglio un testo che - secondo me - rappresenta una delle pietre miliari di provvedimenti legislativi di tutta questa legislatura. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Nicita. nasce diverso tempo fa da una discussione avviata nei Governi precedenti - come hanno ricordato i relatori - coinvolge diverse istituzioni internazionali (in particolare l'OCSE) e il MEF con il Libro verde, esaminando il punto di partenza del nostro Paese nell'ambito della competitività in generale, e poi dalla competitività dei capitali in particolare, che

le specificità europee, e infatti l'Europa è impegnata da diversi anni in tutta una serie di iniziative - alcune delle quali sono ancora in corso - che cercano di completare quella gamba della libertà della circolazione dei dei capitali che è uno dei pezzi importanti e determinanti del *single market*, del mercato unico. C'è infatti un problema di armonizzazione e di competitività dei mercati europei rispetto a quelli internazionali; c'è una specializzazione finanziaria in corso, ma c'è anche la necessità come pure è stato ricordato - di attribuire a questi mercati in tutta l'Europa certezza, sicurezza, tutela dei risparmiatori, indipendenza delle autorità, nonché capacità di promuovere una armonizzazione europea che incrementi non solo la competitività dei singoli Stati membri rispetto agli altri in Europa, ma anche e soprattutto la competitività europea nel quadro internazionale. I punti di partenza sono noti sono stati citati anche recentemente nella relazione di accompagnamento. Rispetto ai dati di qualche anno fa, avevamo una media di quattro società quotate in borsa nel mercato regolamentato italiano; come media annuale è davvero poco. Il 90 per cento delle obbligazioni societarie viene quotato in borse estere e solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali ad azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane. Dall'altra parte, però, gli investitori italiani, sia direttamente che indirettamente, hanno allocato 190 miliardi di euro di euro in *equity*, in investimenti in capitale di rischio oltreconfine. Questo ci dà un quadro della necessità dell'intervento ed è il motivo per il quale il Partito Democratico ma anche le altre forze, partendo dai Governi precedenti, hanno posto il tema della che deve essere data al mercato dei capitali e a tutta una serie di riforme che vanno fatte e riguardano la trasparenza, l'educazione finanziaria, l'indipendenza delle autorità di vigilanza e anche alcuni strumenti di *governance*. A tale proposito mi piace richiamare una notizia positiva che è contenuta nell'ultimo rapporto dell'OCSE, secondo cui in realtà le piccole e medie imprese italiane hanno

entrare nel mercato dei capitali e ravvivarlo, in effetti costituiscono una domanda potenziale molto interessante. Venendo alla questione della riforma e quindi di come noi stiamo intervenendo, devo dire che siamo partiti da un testo che abbiamo ereditato dai Governi precedenti e che affrontava con equilibrio alcune questioni; naturalmente abbiamo una diversa coloritura su alcuni punti in particolare, ma il quadro e l'impianto complessivo erano condivisibili ed erano quelli da cui siamo partiti, con alcuni pilastri fondamentali: certezza, trasparenza, semplificazione, in particolare semplificazione nell'accesso al mercato dei capitali; cito anche la questione della *governance* andando a ridefinire alcune questioni di equilibrio della *governance*, la disciplina

prima ancora che nel merito, ha visto a un certo punto perdere l'impostazione di equilibrio che era stata data. Quando affrontiamo questi temi - mi riferisco soprattutto alla *governance* - dobbiamo tenere presente innanzitutto che le esigenze degli investitori e dei finanziatori devono contemperare contemperare diversi portatori di interesse; quando parliamo di conflitti di interesse fra *management* e azionisti, dobbiamo tenere presente che esistono ovviamente dei modelli internazionali ai quali noi vogliamo convergere, che vanno però poi trapiantati nella specificità dei capitalismi, della *diversity of capitalism* che ciascun Paese ha anche come tradizione. Quindi noi qui abbiamo da contemperare un *trade-off* abbastanza evidente e difficile, che ha bisogno di equilibrio, tra quella che è l'esigenza del *management* di poter avere la libertà ed esprimere la propria azione e quella degli azionisti che devono tutelare i propri investimenti. Nel far ciò vanno evitati due rischi opposti: da una parte, quello che viene chiamato *short termism*, cioè la speculazione, l'ingresso di investitori che semplicemente fanno quello che si chiama *hit and run*, "prendi i soldi e scappa", senza investimenti di lungo periodo, soprattutto in alcuni settori strategici; dall'altra parte, però dobbiamo evitare il rischio dello *status quo*, situazioni cioè nelle quali anche le riforme di *governance* di fatto bloccano in una situazione statica quella che è la dinamica delle società. Si verrebbe così a perdere un punto fondamentale del mercato per il controllo delle imprese, cioè l'idea che il potenziale investitore, che vuole entrare in un'azienda perché convinto di poter portare un valore aggiuntivo, abbia invece una deterrenza perché ritiene che le regole siano talmente asfittiche da non poter portare il proprio contributo di pungolo a quelli che sono i progetti della società. Il punto di partenza era un punto di equilibrio; c'è stata poi una sorta di caotica rincorsa, in particolare sui punti che riguardano il voto maggiorato e plurimo. Era un'esigenza che vi era ed era stata tracciata già nel Libro verde del MEF, dove sostanzialmente si chiedeva un punto importante: l'armonizzazione anche su questo tema, perché abbiamo diverse imprese che poi, alla fine, vanno a cercare altrove la propria collocazione e la propria scelta finanziaria in funzione di queste tipologie di garanzia. Rispetto ad alcune

voto plurimo e maggiorato per poter far valere il proprio investimento, anche rispetto a un rischio che esiste di liste del CDA che possono essere bloccate o riproporre tutte insieme persone da nominare in un'unica lista senza la possibilità di avere una sorta di flessibilità e con un rischio di *status quo* e di troppa vicinanza al *management*, e - dall'altra parte - per evitare il rischio che non ci siano più un orientamento, una proporzione a quel principio *one share*, *one vote* che comunque alla fine è il meccanismo di liquidità e di segnalazione di efficienza del mercato dei capitali. Ci sembra che, rispetto ad alcune proposte che perdevano di vista l'equilibrio, si sia poi alla fine fatto un tentativo da parte del Governo, nel dialogo con la sua maggioranza, che noi abbiamo stimolato anche con le nostre osservazioni. C'è però un punto di fondo: sostanzialmente su questo tema si ritorna

poi alla fine il Governo ha indicato la possibilità di una delega su questo per andare a reintervenire sul TUF. Rispetto a questo dibattito la questione che a noi pare dirimente è che va bene un percorso di delega, ma non ci può essere una delega in bianco. Noi abbiamo indicato, restando abbastanza colpiti dal fatto che non sia stato accettato, un comitato tecnico - come si fece comitato tecnico - come si fece per la riforma del TUF anni fa - di tecnici ed esperti perché la materia è complessa e noi alla fine dobbiamo portare un equilibrio istituzionale che vada bene per tutto il Paese in una prospettiva di crescita. circostanza per la quale il Governo non ha accolto questo comitato noi la riteniamo abbastanza grave perché, come ha dimostrato il dibattito nella Commissione, il Governo, con la propria maggioranza, molto spesso, su temi complicati e complessi, non riesce a tirar fuori il meglio possibile per il Paese. Noi ci siamo stati e siamo in Commissione per questo, ma riteniamo che riforme così importanti

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, l'esigenza di utilizzare meglio e bene i mercati - lo ha ricordato prima il senatore Nicita - per rafforzare e aumentare la capitalizzazione delle imprese resta purtroppo, anche dopo questo provvedimento, un tema di straordinaria attualità, una necessità. Noi sappiamo perfettamente che l'ossatura imprenditoriale del nostro Paese è composta da medie e piccole imprese, che devono senza dubbio trovare nei mercati ambiti e spazi per capitalizzarsi meglio, condizione fondamentale per un accesso al credito composto, composto, ordinato e finalizzato soprattutto ad interpretare i cambiamenti che, nell'economia e nella società, attraversano un modello di sviluppo che deve inevitabilmente essere nuovo, senza gli investimenti delle imprese e senza un utilizzo pieno dei mercati in questa direzione, il tema della bassa capitalizzazione delle piccole e medie imprese resta una questione fondamentale da affrontare. Lo dico con chiarezza: ho ascoltato le relazioni del senatore Damiani e del senatore Orsomarso, ma continuo a considerare l'iniziativa del Governo insufficiente e inadeguata, senza una visione dello sviluppo economico. Continuo a pensare che un tema come questo poteva essere un'occasione straordinaria per aumentare la tracciabilità delle operazioni, per rendere al mercato la fiducia necessaria per investire nelle medie imprese. In questo Paese l'elemento della fiducia resta una delle grandi questioni attualmente irrisolte, anzi, io continuo a dire che vi è la confusione di un Governo che mi sembra più orientato ad autocelebrarsi o a fare opposizione al passato piuttosto che ad affrontare il terreno fondamentale della crescita economica. Siamo di Siamo di fronte ad un intervento riparatorio e di equilibrio del Governo, che si è reso necessario per evidenti, disomogenee complicazioni e diversità di intervento da parte della maggioranza di Governo. Infatti si è agito con emendamenti spesso confusi, improvvisati, quasi tali da compromettere l'equilibrio fondamentale che lascia inevitabilmente agli statuti delle aziende quotate l'elemento fondamentale per definire la *governance*. Attenzione: quando la politica mette mano alla *governance*

con un emendamento. In poche parole, avete costretto il Governo, di fronte a posizioni molto diverse tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, a introdurre in una delega ad un collegato, una delega in bianco per una riforma, peraltro in bianco, del testo unico che - non dobbiamo dimenticarlo mai - fu frutto di un lavoro importante a fronte di un dibattito vero nel Paese tra capitali, associazioni, economisti e autorità preposte competenti. Ci avete chiesto una delega in bianco per una mediazione che non c'è stata, a fronte di un provvedimento che ha trovato nel Governo, anziché la voglia di governare il Paese e di avere una visione per lo sviluppo economico, la voglia di celebrare le divisioni interne alla maggioranza. Ora, voi capite che c'è una distanza enorme tra quello che state comunicando in termini celebrativi dei risultati ottenuti in quest'anno di Governo, di fronte ad un'esigenza che noi comprendiamo e che condividiamo; c'è bisogno di allineare ai Paesi più importanti d'Europa anche le regole fondamentali del rapporto con i mercati del nostro Paese. a quello che avete combinato dentro questa approvazione in quest'Aula oggi, credo che ci siano di mezzo un dilettantismo, un'improvvisazione e una confusione insostenibili per lo sviluppo economico di questo Paese. È il motivo principale per il quale il Partito Democratico vi aveva presentato emendamenti che tentavano di dare a questo punto contenuti tecnici ed economici, con autorità competenti, per aprire un vero dibattito tra economisti, in una relazione con la società e i mercati, se vogliamo fare una vera riforma del testo unico. Invece oggi vi siete presentati in quest'Aula con una delega sostanzialmente in bianco, senza alcun progetto, senza alcuna visione. Io non ho ascoltato l'obiettivo di Governo da parte dei relatori in quest'Aula; non l'ho compreso e me ne scuso. Ho grande rispetto della vostra capacità e della vostra competenza; tuttavia, credo che non si sia compreso, perché è totalmente assente, da parte del Governo, un'idea dello sviluppo economico, della crescita e soprattutto del rafforzamento della dorsale fondamentale delle medie e piccole imprese, che saranno decisive per la competitività economica e per generare nuova e buona occupazione. Questo per noi è il punto più importante dal quale dovete ripartire. Mettete via l'autocelebrazione, cominciate a governare il Paese di fronte ad una responsabilità che avete, quella di guidare la crescita economica. Non troviamo alcuna misura utile per la crescita in questo anno di Governo.

è l'ulteriore dimostrazione. Cambiate strada e fatelo in fretta; dobbiamo guardare alla crescita, perché la crescita economica dovrà determinare nuova e buona occupazione.

che oggi discutiamo e che fa parte degli allegati alle decisioni di bilancio è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Per portare avanti questa riforma il Governo ha fatto un ottimo lavoro di sintesi, con riferimento anche ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi. Infatti, nel marzo 2022 il MEF ha pubblicato un libro verde sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, in cui si sottolineava come la piazza italiana dei capitali manifesti una condizione di cronico ritardo rispetto a quella delle altre economie avanzate, a causa di debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento e per la presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. and development (OECD) Capital market review of Italy for 2020, pubblicato dall'OCSE, ci si interrogava su come creare opportunità di crescita per le imprese e i risparmiatori italiani e si segnalava che nel corso degli ultimi dieci anni una media inferiore a quattro società all'anno è stata quotata sul mercato regolamentato dalla borsa italiana, mentre la capitalizzazione del mercato del Paese in percentuale al PIL si era attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Grazie al Governo Meloni, abbiamo finalmente un testo di legge che mira a dare risposte a questi problemi, in maniera organica, per portare l'Italia su un campo più competitivo a livello internazionale. Prima di addentrarmi nei dettagli del disegno di legge n. 674, vorrei parlare dell'articolo che ritengo di più grande rilevanza nell'ottica della crescita sociale ed economica della nostra Nazione. Finalmente, con l'articolo 21 si parla di partecipazione piena e consapevole dei cittadini italiani alla vita economica del Paese. Finalmente, MEF e Miur sono incaricati di elaborare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il mio personale auspicio è che il Governo riesca a supportare, con una dose di risorse più consistenti, questa bellissima decisione. Finalmente, con questo disegno di legge si riconosce il diritto alla formazione economica e finanziaria, prima lasciata all'iniziativa di singoli istituti scolastici o associazioni, e la si inserisce come insegnamento nelle ore di educazione civica per dare una prima conoscenza ai nostri ragazzi di finanza personale, di risparmio, di investimento e di finanza digitale e dematerializzata. L'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria è ormai riconosciuta a livello internazionale: possedere a livello individuale competenze utili per compiere scelte economiche in maniera responsabile e consapevole accresce il benessere economico delle persone e risulta una condizione fondamentale non solo per l'inclusione finanziaria, ma anche per quella sociale, perché sviluppa maggiore capacità di autotutela e consapevolezza. Per il futuro delle nuove generazioni è importante che questo insegnamento abbia trovato il suo campo di applicabilità nella scuola, perché essa è la struttura educativa maggiormente deputata a far acquisire progressivamente le competenze ai futuri cittadini, con il fine di compiere in modo consapevole scelte - e, nello specifico, scelte finanziarie - adeguate alle proprie esigenze e possibilità. Oggi è inevitabile doversi confrontare con molteplici e frequenti decisioni in questo campo, dall'utilizzo dei pagamenti elettronici alla richiesta di un mutuo, passando attraverso la programmazione pensionistica. Di contro, le statistiche ci mostrano che su questo gli italiani hanno competenze finanziarie ridotte e inferiori, se rapportate a quelle dei cittadini di altre Nazioni. I fattori culturali sono quelli che ne hanno determinato il peso maggiore e pertanto, a chi pone dubbi sul fatto che l'educazione finanziaria debba essere introdotta a scuola alla luce del contesto attuale, riteniamo che la risposta debba essere significativamente «sì». Per fortuna, l'educazione civica è tornata ad essere un insegnamento attualmente obbligatorio e le finalità dell'articolo 21 di questo disegno di legge sono esattamente in linea con la legge istitutiva della materia, la legge n. Le competenze economiche e finanziarie contribuiscono a sviluppare una cittadinanza attiva e utile e promuovono la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. In secondo luogo, l'inserimento dell'educazione economica e finanziaria in insegnamenti equiparabili a quello italiano dell'educazione civica è una strada intrapresa già in altri Paesi. Sulla base dell'ultimo censimento OCSE, infatti, diverse Nazioni lo hanno introdotto o lo stanno introducendo come insegnamento obbligatorio nella scuola, anche se in maniera eterogenea, a seconda delle differenze del contesto istituzionale e della propria organizzazione scolastica. L'articolo 21 rappresenta pertanto il primo passaggio di un percorso verso la diffusione sempre più strutturata delle tematiche economico-finanziarie tra gli insegnamenti curriculari. È una misura importante e urgente per proseguire con maggiore forza ed efficacia il percorso verso un innalzamento della cultura economica e finanziaria dei giovani. È indubbio, infine, che una maggior conoscenza tra i cittadini di queste materie sul lungo termine aiuterebbe anche il corretto funzionamento dei mercati, dando il suo piccolo, ma importante contributo alla loro stabilità. Venendo alle principali proposte a cui fa riferimento il testo che esaminiamo oggi, esse incidono sulla disciplina delle società di capitali, con l'obiettivo di sviluppare il mercato italiano e renderlo più attrattivo, sia attraverso l'offerta di servizi di investimento più competitivi da parte dell'industria finanziaria nazionale, sia mediante la rimozione di alcuni degli ostacoli alla domanda di capitali da parte delle imprese. Queste misure si pongono inoltre come esigenza indifferibile e condivisa, visto che si inquadrano nell'ambito degli adeguamenti a normative europee provenienti da Bruxelles, tendendo, da un lato, a rimuovere o attenuare vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza sul mercato da parte delle imprese e, dall'altro, indirizzando gli investimenti verso il tessuto produttivo e semplificando alcune previsioni in materia di intermediari. L'approvazione di questo disegno di legge pertanto è un obiettivo ambizioso, urgente e indispensabile per l'economia del Paese. Il disegno di legge per la competitività dei capitali si propone come un pacchetto di interventi organico, che mira a incentivare le quotazioni delle società e a diffondere l'azionariato della borsa italiana. Il provvedimento contiene modifiche al testo unico della finanza, al codice civile e ad alcuni decreti adottati nel pieno della crisi Covid introduce semplificazioni normative e operative volte a facilitare il ricorso delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, al mercato dei capitali e in alternativa al solo mercato tradizionale del credito per realizzare i nostri obiettivi di crescita. Questo provvedimento si inserisce in un contesto di progressivo rafforzamento della struttura finanziaria, intrapreso dalle aziende italiane nell'ultimo decennio, accompagnandole verso una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, realizzata attraverso l'emissione di titoli obbligazionari e l'aumento di nuove quotazioni in borsa. Tutto ciò va nell'ottica di contribuire a ridurre la dipendenza delle aziende dal credito bancario, particolarmente diffusa fra le Infatti, per le imprese di minore dimensione l'accesso al finanziamento alternativo è ostacolato da rilevanti barriere all'entrata. In particolare, le emissioni di titoli sono contenute a causa degli elevati costi fissi unitari delle operazioni e del minore interesse degli investitori con imprese con bilanci ovviamente di di norma più rischiosi. Sono perciò evidenti i benefici che un mercato di capitali sviluppato può portare all'economia di un Paese: da un lato, consente alle imprese una riduzione del costo di capitale e crea una sana diversificazione delle fonti; dall'altro, il confronto e l'interlocuzione costanti con investitori istituzionali, nazionali e internazionali offre opportunità interessanti, come lo sviluppo del *business*, il rafforzamento della *governance* dei fattori ESG e, in generale, opportunità di crescita e sviluppo. con questo disegno di legge il Governo Meloni ha voluto avviare un vero e proprio cambio di passo strutturale nel rapporto tra imprese e mercato dei capitali, da un lato, rimuovendo vincoli normativi e operativi modificando l'accesso al mercato da parte delle imprese e, dall'altro, ancora introducendo misure che stimolano, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti attraverso i mercati. Non ultimo e non meno importante, il Governo Meloni si è occupato anche di una forma di investimento che indubbiamente è la più importante, cari colleghi: il capitale umano, capace di generare nel prossimo futuro una conoscenza finanziaria che possa apportare implicazioni in termini di benessere individuale e sociale per affermare un cambiamento fondamentale della nostra Nazione.

grande emozione per quello che all'epoca era il cuore della crescita dell'Italia degli anni Ottanta perché era il luogo in cui il risparmio degli italiani aveva trovato un nuovo impiego, dopo essere stato mobilitato per la prima volta Il passaggio era stato, direi, naturale: dai titoli di Stato ci si era mossi sui fondi di investimento e, indirettamente o direttamente, quindi dai fondi di investimento o dal risparmio diretto, alla Borsa. quindi, come luogo fisico di mercato, non sarebbe durata molto, perché di lì a poco, dai primi anni Novanta, il mercato diventò telematico

per cercare di riprendere in mano la competitività del possesso dei luoghi del mercato, perché non è indifferente se il mercato è in Italia o da qualsiasi altra parte nel mondo. Troppo spesso si è temuto o si è creduto che vedere sullo stesso schermo le contrattazioni di diversi prodotti finanziari comportasse che il luogo di scambio fosse lo schermo, così: qualche mercato - si pensi per esempio a quelli iper rischiosi e non regolati sulle criptovalute - era non si sa dove, mentre alcuni altri erano profondamente regolati. Il fatto di riuscire a creare uno spazio di mercato competitivo per le aziende è fondamentale, sia per la crescita delle imprese italiane, sia per la sicurezza degli investitori. In particolar modo vorrei ricordare che al momento le dimensioni della nostra Borsa non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che dovrebbe avere un'economia delle nostre dimensioni. Si pensi che alcune delle principali aziende italiane hanno scelto di non quotarsi: cito, per esempio, i casi Ferrero o Barilla, per dire nomi conosciuti da tutti, che sono aziende di enorme importanza sia strategica sia occupazionale per l'Italia, che hanno deciso da sempre di non quotarsi, non trovando attraente la possibilità di raccogliere capitali nei mercati finanziari e nella Borsa. sono state ritirate dalla quotazione in tempi non sospetti, invece altre ancora hanno deciso di quotarsi altrove, tipicamente in luoghi dove magari la regolamentazione era più competitiva, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista delle delle regole: un caso tipico, per esempio, è quello dell'Olanda, che in certi frangenti agisce in modo predatorio nei confronti degli altri Paesi; tuttavia, se c'è un predatore, dall'altra parte non bisogna farsi preda, per cui bisogna cercare, per quanto possibile, di adeguare le nostre regole in modo tale da rendere un ecosistema competitivo, per far sì che le nostre aziende continuino a fiorire in un mercato nostro. Anche l'acquisizione di Borsa italiana da parte del London stock exchange è stata oggetto di diverse tappe che hanno portato poi a soluzioni di compromesso e che tuttora in futuro potrebbero portare a modifiche, ma tutto dev'essere subordinato a una regolamentazione precisa del nostro approccio ai mercati dei capitali.

Quante volte abbiamo visto pubblicità molto invasive, in tempi recenti, di strumenti che propagandavano cose che sembravano azioni, ma che in realtà non lo erano? Ho fatto anche le mie segnalazioni, perché in certi casi mi mettevo nei panni di un consumatore o di un risparmiatore non particolarmente esperto in questioni di mercati derivati o di prodotti strutturati, potuto avere la precisa sensazione che alcune piattaforme (sempre propagandate con la magica formula del tasso zero, commissioni zero, interessi zero, tutto a zero)

su quelle azioni, in realtà si assumeva il rischio controparte di quella piattaforma del mercato. Il fatto di avere una regolamentazione precisa su questi temi è un primo passo per quello che mi auguro diventerà un grande mercato dei capitali, che potrà aiutare la futura crescita dell'Italia.

migliorare alcune norme di semplificazione, il correlatore nel suo intervento precedente ha ricordato la possibilità di intervenire

una metafora che ha utilizzato il ministro Crosetto. Noi oggi abbiamo di fronte una montagna: per scalare una montagna o ti impressioni e non l'affronti per nulla o devi cominciare a puntellare. Questo provvedimento arriva anche da altri Governi e noi abbiamo provato a

sottolineare che un settore di imprese italiane (ad esempio, Barilla o Ferrero), di genio italico e di grande operosità italiana, ha deciso di non stare nella turbolenza dei mercati, in cui spesso le speculazioni e altro hanno rappresentato una grande rottura. In Commissione abbiamo ascoltato un pezzo di capitale italiano tipico della struttura di questo nostro Paese, che ha dentro 11 miliardi, e che non vuole fare il passacarte, ma avere un sistema di *governance* che tenga conto anche di queste ragioni. Questo è il metodo, questo il merito. Rispetto a tutte le altre questioni,

fiscale ed a un sistema di *compliance* che guarda alle nostre imprese non come a un nemico da battere, da tassare e stratassare, ma da accompagnare insieme a un nuovo mercato di capitali, con banche magari governate con il principio del merito (e, anche lì, il metodo: chi decide?). Queste sono in sintesi le motivazioni che ci hanno

quasi ogni anno. Questa è la sintesi degli interventi. Non abbiamo trattato la questione con sufficienza, ma abbiamo fatto una relazione avendo lavorato molti mesi e penso che tutta l'Assemblea, compresa la minoranza, non meriti mai l'atteggiamento della sufficienza o della presunzione.

Credo che, se avessimo chiesto a un ignoto passante conoscitore del mercato finanziario fino a un anno fa di dirci qual era lo stato di salute del mercato finanziario in Italia, avrebbe potuto rispondere, magari citando Montale, che solo qualcosa ci poteva dire, cioè ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ecco, a distanza di un anno, lo stesso ignoto passante che dovesse trovarsi a guardare l'assetto normativo del mercato dei capitali italiano, certamente troverebbe degli enormi passi avanti.

rispetto alla formulazione con cui è entrato in questo ramo del Parlamento, ne esce certamente accresciuto e migliorato nell'ottica di garantire, sempre e comunque, che la crescita del mercato dei capitali sia omogenea e in linea omogenea e in linea con le prassi di mercato. Non dobbiamo ignorare infatti che il mercato dei capitali non è e non può essere un fenomeno squisitamente domestico, ma assume una rilevanza strutturale soprattutto a livello di interrelazioni sovranazionali. In quest'ottica, In quest'ottica, il Governo ha sottoposto al Parlamento un emendamento, che il Parlamento, almeno in Commissione, ha recepito, che è quello che ci ha portato ad affiancare al disegno di legge capitali nella sua formulazione originaria, come modificata dagli emendamenti,

È una delega, e lo dico anche per tranquillizzare l'opposizione, che il Governo non intende esercitare in autonomia, chiuso in segrete stanze, senza coinvolgere gli esperti. Personalmente, e a nome del Governo, do per scontato che il testo del decreto delegato sarà collazionato col supporto degli esperti e che, quando il Parlamento darà il proprio contributo alla revisione di quel testo, lo farà col supporto degli esperti. È un testo, quello della delega, che porterà il mercato dei capitali italiano a fare un ulteriore passo avanti; un passo avanti che dovrebbe, per lo meno nelle intenzioni, condurre il nostro mercato dei capitali ai livelli di quelli europei, non per capitalizzazione probabilmente - ci vorrà qualche anno - ma certamente per impatto regolatorio, perché un mercato dei capitali funzionante è un mercato di capitali che ha un impatto regolatorio affidabile, perché si investe su un mercato quando quel mercato viene ritenuto affidabile. Il sistema Paese è affidabile e il mercato dei capitali italiano diventerà pienamente affidabile grazie all'implementazione che questo disegno di legge e la successiva delega daranno al mercato dei capitali. Ringrazio dunque

miglioramento del testo base portato dal Governo in questo ramo del Parlamento. Grazie ancora a tutti voi, con l'auspicio di poterci ritrovare a breve per dire esattamente ciò che siamo e ciò che vogliamo del mercato dei capitali.

con riferimento a questo emendamento, il MoVimento 5 Stelle chiede la possibilità di apportare una modifica all'articolo 2389 del codice civile in tema di determinazione dei compensi dell'organo amministrativo. È bene che, nel momento in cui c'è una società quotata o una società a partecipazione pubblica a rilevanza sociale, la definizione dei compensi spettanti all'organo amministrativo vedano anche la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti tra particolari figure professionali e di competenza nel settore, in modo tale da favorire l'equità salariale all'interno della stessa società quotata o della stessa società a partecipazione pubblica.

rimettendo allo statuto, secondo ovviamente le indicazioni e le regolamentazioni delle autorità competenti, Consob *in primis*, di far sì che la presentazione della lista avvenga nella modalità più trasparente e più a garanzia delle minoranze possibile, senza intervenire in maniera che noi riteniamo macchinosa e farraginosa

Siamo stati favorevoli, ma andando a stabilire, al contempo, una serie di limiti allo strapotere dell'organo amministrativo, per evitare il rischio di avere organi amministrativi fotocopia che si ripetono nel tempo. Per questo motivo, nell'emendamento oggetto di discussione, proponiamo due limiti importanti. Da una parte, si limita la possibilità che gli amministratori uscenti possano ricoprire il 100 per cento della al 50 per cento dei posti disponibili, in modo tale da favorire il passaggio manageriale a giovani che generalmente sono sinonimo anche di innovazione. Dall'altra parte, poniamo un altro limite allo strapotere dell'organo amministrativo, ponendo fine agli incarichi plurimi in moltitudini di società, anche quotate, così come anche a incarichi che si ripetono all'infinito nel tempo, proponendo un limite massimo di nove anni per la ripresentazione della propria candidatura nell'ambito delle liste del Consiglio

Presidente, sempre in merito al provvedimento sul voto maggiorato, noi siamo favorevoli al voto maggiorato rispetto al voto plurimo, così come peraltro proposto dal Governo, con riferimento alle società quotate. Sul punto, signor Presidente, mentre il Governo propone un voto maggiorato senza porre delle condizioni, delle condizioni, la nostra proposta mira a riconoscere sì un voto maggiorato, condizionandolo però ad un principio che vorrebbe favorire la stabilità finanziaria all'interno delle società quotate. andiamo quindi a prevedere un voto maggiorato, in funzione del tempo di stabilità finanziaria e di possesso delle azioni, a quegli azionisti che dimostrano fedeltà nel possesso delle azioni. delle azioni. Con questo provvedimento chiediamo al Governo di valutare attentamente gli effetti che il voto plurimo può avere sulle nostre società e soprattutto sugli obiettivi del disegno di legge, favorendo invece un voto plurimo, in modo tale da condizionarlo al tempo di possesso dell'azione o del titolo societario e da contrastare anche il fenomeno della speculazione.

poniamo dei limiti, *in primis* al fatto che possano essere poste delle limitazioni alla cessione delle azioni a cui viene attribuita la facoltà di voto plurimo, e poi introduciamo la possibilità di stabilire un lasso temporale entro cui il voto plurimo si può esercitare, quindi non *ad infinitum*, in modo che gli statuti possano prevedere dei periodi di tempo determinati. Ci sembra una misura che contempera diverse esigenze.

al Governo che andare a modificare questo parametro senza condizionarlo al parere vincolante, in base ai trattati europei, della BCE, crea confusione nell'ambito del sistema bancario. Noi oggi siamo andati a modificare una norma senza avere un preventivo parere positivo della BCE. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che questa norma non dice cosa accade a quelle banche popolari che non hanno la possibilità di aumentare l'attivo patrimoniale - attenzione: non è il capitale,

Oggi viviamo in un momento di desertificazione bancaria, dove cittadini e imprese non hanno la possibilità di accesso non solo al credito, ma anche alla moneta bancaria. Ci sono territori, soprattutto nel retroterra, dove lo sportello bancario è un vero e proprio miraggio. E con questa norma non favorite il contrasto alla desertificazione.

Signor Presidente, anche di questo tema si è parlato in discussione generale. Semplicemente, noi chiedevamo la costituzione di una commissione tecnica, composta da esperti di alto profilo internazionale, che accompagnasse il Governo nell'attuazione della delega, soprattutto in riferimento alle tematiche maggiormente tecniche. in Commissione questo emendamento è stato respinto. Ricordo che la delega fiscale prevede la composizione di una commissione tecnica per accompagnare il Governo nell'attuazione Non capiamo perché, invece, su questa materia non si possa mettere nero su bianco che il Governo, su alcune tematiche di rilievo internazionale, dall'alto contenuto tecnico, si faccia accompagnare da esperti indipendenti sulla materia.

Sempre con riferimento all'articolo 16-*ter*, andiamo a riproporre una norma che stiamo riproponendo da diverso tempo, già dalla scorsa legislatura, che si ispira al pensiero di Adriano Olivetti: Olivetti: favorire il rapporto di equità salariale tra il *manager* e l'ultimo dei lavoratori stipendiati all'interno delle società, soprattutto di quelle quotate, in modo tale da garantire questo rapporto nel tempo, senza favorire solo l'aumento salariale del *manager* a discapito della forza lavoro. Proponiamo quindi che questo rapporto venga mantenuto nel tempo da 1 a 50. 50. In ultimo, Presidente, sempre con riferimento al limite allo strapotere dell'organo amministrativo, proponiamo un limite ai mandati sia dell'organo amministrativo sia degli organi di controllo

nei controlli societari.

(lo rileggo): «sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi», con l'inserimento quindi delle parole

Noi qui abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione, grazie anche alle aperture del Governo, perché nella prima formulazione si parlava solo di educazione finanziaria,

relatori e il Governo - anche l'inserimento del riconoscimento della cultura di fare impresa. Oggi, per raggiungere l'obiettivo della competitività dei capitali e e della crescita economica dell'impresa, non basta regolamentare semplicemente al meglio il mercato finanziario; per raggiungere questo obiettivo occorre aiutare

È stato un lavoro intenso quello fatto in Commissione e probabilmente è una delle prime volte che accade per un provvedimento di questo genere: abbiamo avuto il tempo necessario per farlo, anche perché è stato fatto con una collaborazione forte anche da parte dell'opposizione. Questo fa Questo fa capire che, quando si vuole, si riescono ad ottenere risultati importanti in termini di regolamentazione. È un provvedimento che probabilmente tocca poco nell'intimo gli italiani

ad avvicinarla ad altri mercati che hanno una tradizione molto più vasta rispetto alla nostra e regolamentata in maniera completamente diversa. Unitamente a questo, c'è anche una delega al Governo che farà crescere ancora di più questo provvedimento. Com'è stato dimostrato in questi in questi giorni di lavoro, il Governo ha detto che non avocherà a sé esclusivamente la stesura dei prossimi provvedimenti, ma li vedrà insieme a noi in Commissione. molto importante, che adeguerà l'Italia da un punto di vista regolamentare, in modo tale che il mercato finanziario in Italia possa diventare molto più attrattivo e tutelare gli investitori:

Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, il nostro intervento sarà limitato al tema dell'educazione finanziaria. Dall'ultima indagine triennale della Banca d'Italia emerge un'obiettiva vulnerabilità degli italiani a errori e truffe e questo perché l'educazione finanziaria in Italia non non ha raggiunto un livello soddisfacente, né sufficiente per mettere al riparo i cittadini e le cittadine da scelte sbagliate, da costi eccessivi e, appunto, da truffe. L'indagine in questione parla

Da questi dati risulta chiaro il bisogno di investire nell'educazione finanziaria. L'accordo sottoscritto fra l'università di Bolzano e la Banca d'Italia, proprio per creare percorsi mirati per gli studenti di Scienze della formazione, che come futuri insegnanti avranno la possibilità di far conoscere anche ai più piccoli gli strumenti capaci di favorire autonomia e scelte responsabili di consumo e di spesa, va in questa direzione. allora sicuramente positive le norme contenute in questo provvedimento, che portano l'educazione finanziaria all'interno degli insegnamenti di educazione civica nelle scuole, come elemento per la partecipazione piena e consapevole alla vita economica. È importante che tutto questo sia all'interno di un provvedimento pensato per accrescere la competitività italiana e il sostegno all'economia, con l'obiettivo di promuovere interventi di ammodernamento del quadro normativo, alla luce delle delle dinamiche evolutive dei mercati e della crescente concorrenza tra piazze finanziarie internazionali. Questa misura, come specifica la Banca d'Italia, è inserita in un contesto di progressivo rafforzamento della struttura finanziaria intrapreso dalle imprese italiane nell'ultimo decennio e, da un lato, tende a rimuovere o ad attenuare vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza nel mercato da parte delle imprese, dall'altro, a indirizzare gli investimenti verso il tessuto produttivo, semplificando alcune previsioni in materia di intermediari. Nonostante questi sviluppi positivi, il divario tra la dimensione dei mercati dei capitali italiani e quella dei principali Paesi europei resta però Fra le ragioni di queste differenze vi sono la limitata dimensione media delle aziende quotate italiane e la minore propensione ad accedere al mercato. Proprio quest'ultimo aspetto, dal nostro punto di vista, è fondamentale per comprendere la reale e fattiva importanza dell'educazione finanziaria, una formazione di base più efficiente contribuirebbe a un cambio di passo interessante nella competitività del mercato italiano. Cittadini che meglio conoscono la finanza e il funzionamento dell'economia non sono solo cittadini che gestiscono meglio le loro finanze, ma sono anche cittadini che hanno maggiori strumenti per comprendere il funzionamento della finanza pubblica e quindi per valutare le scelte compiute in sede politica. L'inserimento dell'educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado può darci una marcia in più per comprendere le dinamiche socioeconomiche che ci circondano e, in un mondo che va avanti velocemente, come Paese dobbiamo essere in grado di concedere nuovi strumenti alle giovani generazioni e di creare sempre più opportunità al passo con i tempi.

non abbiamo potuto seguire direttamente la discussione in merito al provvedimento, ma vorrei sottolineare alcuni aspetti, partendo da un dato. Questo provvedimento negli intenti era considerato un fatto di grande positività, perché interviene in particolare nella questione delle piccole e medie imprese. Devo dire, però, che oggettivamente, al risultato finale, sono più le ombre delle luci. Sottolineo subito che noi ci asterremo su questo provvedimento, proprio per queste ombre. Vorrei sottolineare, in particolare, la questione delle piccole e medie imprese. Discutiamo certamente di società di capitali,

cioè avere un sistema in cui ci sono servizi a livello del territorio, una produzione e una formazione della manodopera, una capacità di unirsi per intervenire sui mercati internazionali e un sistema di credito. Per questo è nato in passato un sistema di banche

soprattutto salvaguardare il sistema, la rete, cioè questo tessuto distributivo nel territorio che vada in tale direzione. Non è solo un atto del Novecento, perché anche in questo periodo, anche nelle migliori famiglie, accade questo. Invece voi avete introdotto una

ho già posto questo problema in passato, ma se un'impresa ha un compito sociale, è chiaro che si deve fare carico delle difficoltà:

non solo alla capacità di conoscere la previdenza e a tutto ciò che bisogna fare, ma soprattutto al fatto che ha anche una responsabilità sociale. Per questa ragione, per queste lacune che ci sono e che ho cercato di sottolineare, pur brevemente, noi ci asterremo sul provvedimento in

una serie di disposizioni che erano molto attese da quasi tutti gli *stakeholder* e gli operatori finanziari. Si tratta di diverse norme che, a vario titolo, costituiscono un intervento importante in materia finanziaria e che, ne siamo certi, consentiranno il rafforzamento della competitività del nostro sistema e una maggiore apertura del mercato alle piccole e medie imprese, nell'ottica, da un lato, di favorirle, attraverso la quotazione e il rafforzamento patrimoniale, dall'altro, di consentire loro nuove forme di finanziamento che prescindono, almeno in parte, da quello squisitamente bancario. Le nostre imprese, durante i periodi di crisi, sono state investite e hanno sofferto maggiormente rispetto alle loro cugine d'oltralpe e di oltremanica, perché piccole e ancora poco integrate nel sistema produttivo europeo; perché fatte ancora di singole eccellenze, frutto dell'inventiva e del coraggio dei nostri imprenditori, ma non appieno parte della filiera del nostro continente; perché vivono, anche se meno di un tempo, dei finanziamenti del credito bancario, prive o quasi di strumenti finanziari che consentano una capitalizzazione alternativa. Una vera competitività dei mercati finanziari e dei capitali interessa anche le banche, tanto come emittenti, in quanto le banche sono tra le principali società quotate ed emittenti di strumenti finanziari (ad esempio, titoli obbligazionari) con i quali raccolgono risorse per supportare al meglio l'economia reale, quanto come consulenti, in quanto le banche supportano le imprese ad accedere al mercato dei capitali, tramite attività di ricerca (cosiddetto *scouting*), consulenza (cosiddetto *advisory*), strutturazione e collocamento dei titoli emessi dalle imprese, ma anche e soprattutto come intermediari, in quanto sono gli istituti di credito che contribuiscono all'allocazione del risparmio, essendo i principali distributori di prodotti finanziari e di investimento e consentono agli investitori, soprattutto *retail*, di accedere al mercato in maniera assistita e tutelata. erano quindi assolutamente necessarie e non più rinviabili. Infatti, se guardiamo i dati dei nostri mercati azionari, nel 2022 complessivamente si sono registrate 30 nuove ammissioni (erano 49 nel 2021). Anche se è una proporzione più ampia rispetto a quella di altri Paesi europei, questo dato comunque non è positivo. Il fenomeno più rilevante, oltre al numero ridotto di nuove quotazioni in un anno (da circa dieci anni il numero è inferiore a cinque), è rappresentato anche per l'Italia dalle numerose uscite dal listino. Le condizioni macroeconomiche in cui operano le imprese italiane sono note e le abbiamo accennate, ma ancora più grave è il livello d'incertezza relativamente alle prospettive future: guerra, forniture di materie prime e mercati di sbocco, inflazione e restrizione del credito, disponibilità di manodopera e regime fiscale. In questo quadro, non può stupire che si constatino il preoccupante fenomeno di una certa ritrosia da parte di molte imprese nazionali a quotarsi e il frequente abbandono di molte di esse. Contemporaneamente, si assiste alla fuga di un numero non elevato, ma significativo soprattutto per dimensioni e qualità, di aziende per trasferire le loro quotazioni all'estero, in Paesi - a loro dire - più ospitali. In sostanza, la Borsa in Italia rappresenta sempre meno - basta osservare il decrescente livello della sua capitalizzazione in rapporto al PIL - il volto del capitalismo di successo. Verrebbe da domandarsi se per un'impresa italiana quotarsi in Borsa e in Italia sia ancora considerato essenziale. A livello europeo, queste nuove norme sono complementari e vanno nella direzione del nuovo piano d'azione europeo per l'unione del mercato dei capitali. In Europa i mercati finanziari nazionali sono frammentati e vi sono ampie divergenze tra di essi. Come abbiamo detto, quindi, esistono piazze più sviluppate, a maggiore vocazione internazionale caratterizzate da un ambiente più favorevole alla quotazione e da un'ampia presenza di liquidità e di investitori istituzionali. È fondamentale sostenere la realizzazione dell'unione del mercato dei capitali europeo: penso alle iniziative della federazione bancaria europea, al progetto Markets4Europe, che cerca e propone soluzioni per lo sviluppo e l'integrazione dei mercati di capitali in Europa. Occorre una forte accelerazione a tutte queste norme, che vanno nella giusta direzione. Parlando poi delle modifiche operate nella Commissione di merito in sede referente, bisogna valutare positivamente il lavoro svolto. Non c'è dubbio che il disegno di legge sia stato migliorato: sono state riviste e meglio precisate alcune norme sulla semplificazione in materia di accesso ai mercati di capitali e su alcuni temi che riguardano la disciplina degli degli emittenti di strumenti finanziari diffusi, oltre che sul tema della sottoscrizione delle obbligazioni emesse da società per azioni e dei titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (quest'ultimo è un tema assai delicato, le cui conseguenze vanno spesso a impattare direttamente sui piccoli investitori). Assai positivo poi è il giudizio sull'articolo 16-*ter* introdotto in sede referente, con il quale si delega il Governo ad avviare la revisione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, in particolare al fine di sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, facilitare il passaggio della quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati e, infine, rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a maggior tutela degli investitori. Sull'articolo 16-*bis*, anch'esso introdotto da un emendamento in Commissione in sede referente, invece non possiamo trovarci d'accordo. Riteniamo pericoloso un innalzamento del limite dell'attivo delle banche popolari. Tra l'altro, tale innalzamento è di fatto un raddoppio. Si passa da 8 a 16 miliardi di euro: davvero troppo. Nel 2015 ero alla Camera dei deputati e, proprio in Commissione finanze, affrontammo una serie di crisi bancarie senza precedenti in Italia. A mio avviso, abbiamo messo in sicurezza il sistema bancario, varando le riforme degli istituti di credito cooperativo e delle banche popolari, nel tentativo di preservare il loro rapporto col territorio e, al contempo, di operare con maggiore solidità nel panorama globalizzato. Ora, andare a porre mano a quelle norme, consentendo a banche di dimensioni molto grandi il mantenimento della forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e relativo regime, a nostro avviso

atto un disegno di legge molto articolato per regolamentare il mercato dei capitali, contrariamente a quello che è stato detto fino adesso, cioè che non è stato fatto nulla e che non sono state ascoltate le parti. È un insieme di articoli valutato e scritto con esperti che hanno dato il proprio contributo, dapprima durante la consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e poi, di nuovo, durante l'esame in Commissione finanze al Senato. La Commissione ha svolto un ampio giro di audizioni e raccolto le memorie dei tanti soggetti e associazioni competenti per materia: dalla Consob alla Banca d'Italia, all'associazione delle società quotate, a quelle degli imprenditori, ai grandi studi legali che accompagnano le quotazioni e agli studiosi. Tutti hanno inteso fornire il proprio contributo, che è stato molto prezioso. Si tratta quindi di un testo che ha trovato una larga competenza e convergenza. In Italia il mercato dei capitali ha dimostrato finora di essere assolutamente inadeguato a sostenere la crescita della nostra economia e la spinta pubblica è insufficiente a sostenere un'economia nazionale in rapida evoluzione, anche a causa delle ripetute crisi dei mercati internazionali. Il mercato privato presenta ancora troppi operatori con dimensioni non adeguate e soprattutto non idonee a supportare il lungo ciclo di vita delle aziende, che richiede finanziatori in grado di sostenerne le scelte, delineate dai piani industriali che, come sapete, sono sempre pluriennali. Gli investitori in capitale di rischio, i cosiddetti *venture capitalist*, che in Italia sono presenti, ma ancora di numero ridotto e con propensione al rischio ridotta, spesso accompagnano la nascita e la crescita dimensionale delle imprese fino alla quotazione sul mercato regolamentato. Le quotazioni però sono poche, anzi pochissime, e molti sono i *delisting*, cioè azioni quotate che, dal valore di borsa, non trovano ulteriori stimoli alla propria crescita dimensionale. Per fornire un dato, nel 2022 si sono quotate venti nuove società, per un valore di 4,7 miliardi, ma i *delisting* sono stati venti, per un valore di 43,5 miliardi. L'Italia, ottava potenza industriale al mondo, ha il ventiduesimo mercato regolamentato per valore, con una capitalizzazione di borsa di circa 630 miliardi: meno di un terzo del PIL italiano. Tutti i titoli della borsa italiana valgono meno del 25 per cento del primo titolo quotato a Wall Street, Apple, che vale circa 2.700 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, prima economia del mondo, hanno il primo hanno il primo mercato borsistico al mondo, con un valore di capitalizzazione complessiva di circa 45.000 miliardi di dollari: circa due volte il PIL americano. Parliamo di un mercato borsistico dinamico ed efficiente, quello americano, che attira capitali da tutto il mondo. Altri esempi: la borsa francese vale 2.620 miliardi, pari all'88 per cento del PIL. La borsa olandese vede una capitalizzazione complessiva di oltre 1.080 miliardi, superando il proprio PIL. La borsa olandese ci interessa direttamente, perché, come sappiamo bene, grazie a una regolamentazione molto più favorevole, si è portata via parecchie aziende italiane, quotandole sul mercato di Amsterdam. È aumentato il suo prestigio e il suo giro d'affari. L'apporto di nuovi capitali ha consentito la sua crescita dimensionale e di fatturato, garantendo comunque il controllo degli azionisti di riferimento. Questo disegno legge, tra le altre cose, va nella direzione di rendere più attrattiva l'idea di quotarsi e di rimanere in Italia. Affronta cioè le criticità che frenano le aziende ad entrare in borsa ovvero le inducono ad uscirne, incentivando la quotazione di nuove imprese e facilitando gli aumenti di capitale di quelle già quotate. Il testo affronta complessivamente il tema dello sviluppo dei mercati dei capitali, con misure che favoriscono la raccolta di capitali sul mercato e inizia a rafforzare il ruolo dell'investitore istituzionale nel finanziamento del capitale. Vengono abrogate le norme di regolazione che addirittura eccedevano la previsione della disciplina europea: tra queste, l'obbligo di segnalazione dell'operazione effettuata dagli azionisti di controllo e la responsabilità del collocatore sul prospetto e del controllo di completezza pre-avvio dell'istruttoria di approvazione del prospetto. Viene abolito anche il potere della Consob in materia di obblighi di acquisto e ripristino del flottante per chi venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento del capitale. Ci sono poi una serie di disposizioni che mirano a facilitare le forme di accesso al mercato dei capitali sia nella fase delle quotazioni, che viene semplificata, sia in quella successiva. Viene valorizzata l'autonomia statutaria delle società. In tal senso va la norma, introdotta in Commissione finanze, sulla rappresentanza alle assemblee delle società quotate, che avviene esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società. Le modifiche statutarie, da approvare entro il 2025, regoleranno queste disposizioni. La Commissione finanze ha introdotto un articolo che consente al consiglio di amministrazione uscente di presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione e delle modalità di elezione. Il consiglio di amministrazione approva con la maggioranza di due terzi e propone una lista che contiene il numero dei candidati maggiorato di un terzo; viene rivisto anche il meccanismo di elezione successivo (prima, come sapete, erano quattro quinti). Sono state accolte le norme sul voto plurimo, che diventa estendibile fino a dieci, e, attraverso un nuovo articolo sul voto maggiorato, inserito in Commissione finanze, un meccanismo che darà più potere in assemblea agli azionisti stabili di una società. Ecco perché poi le nostre società avranno più rigore per andare com'è successo per grandi gruppi industriali, perché avremo la possibilità di farlo in Italia. Viene rafforzato il ruolo dell'investitore istituzionale (cioè le casse previdenziali e i fondi di pensione) nel finanziamento del capitale delle società quotate, che in Italia è di gran lunga inferiore a quello del resto d'Europa. Si tratta però di un primo passo, se consideriamo che in Europa la media del patrimonio investito in azioni dagli investitori istituzionali è il 10 per cento, mentre in Italia è fermo all'1 per cento. Si mette mano anche al sistema sanzionatorio e amministrativo della Consob, consentendo di definire il procedimento con modalità negoziali. siamo in presenza di una serie di riforme che avvicinano il modello italiano del mercato dei capitali a quello di altri Paesi europei meno restrittivi e più attrattivi del nostro. L'importante ora è approvare questo testo, che certamente segna una scelta opportuna,

L'ultimo dato della Banca d'Italia, di giovedì scorso, vede un saldo negativo di investimenti italiani all'estero, rispetto a quelli esteri in Italia, di circa 50 miliardi nell'ultimo anno. Gli investitori italiani, anche attraverso i fondi di investimento, hanno quindi spostato i propri soldi all'estero. È necessario che questi capitali rimangano in Italia o vi rientrino e tornino a sostenere l'economia reale italiana. Il testo approvato dalla Commissione finanze include una serie di modifiche ed integrazioni che lo rendono ancora più completo rispetto al testo iniziale. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Nell'ultimo decennio, il nostro mercato dei capitali è stato oggetto di importanti riforme strutturali, volte a migliorare la solidità finanziaria e la dimensione patrimoniale delle imprese. Nonostante le riforme introdotte, esso risulta però ancora formato per circa il 75 per cento da imprese a controllo familiare, con una capitalizzazione di mercato rapportata al PIL notevolmente al di sotto della media europea. Per incentivare la quotazione e la permanenza delle società nel mercato finanziario, si interviene oggi ancora una volta sulla normativa primaria modificando il diritto societario. Prima di entrare nel merito del provvedimento, è doveroso evidenziare che il disegno di legge in discussione risulta in molte parti modificato e migliorato rispetto al provvedimento approvato dal Governo. Si tratta di un'opportunità che in questa legislatura il Parlamento ha avuto solo in rare occasioni. Preliminarmente, mi preme ringraziare il Governo, il presidente Garavaglia, a cui auguro una pronta guarigione, i relatori e tutti i commissari per il lavoro sinergico svolto in Commissione e soprattutto per le attenzioni riservate alle proposte emendative del MoVimento 5 Stelle. Alcune di tali proposte sono state fatte proprie dalla maggioranza e altre, come la soppressione del *quorum* agevolato sugli aumenti di capitale, nonché il provvedimento che estende l'educazione civica anche alla cultura d'impresa e non solo all'educazione finanziaria, oltre alla previsione di obblighi in tema di trasparenza informativa, sono state approvate dalla stessa maggioranza. Tra i temi di particolare importanza ancora da risolvere la dicotomia tra la possibilità concessa alle PMI quotate sotto forma di Srl di accedere a sistemi di dematerializzazione delle quote e l'assenza però di un nuovo sistema normativo adeguato per facilitare il loro accesso al mercato dei capitali. Si conserva infatti lo stesso ordinamento codicistico di un modello di società chiuso, focalizzato sulla persona del socio più che sulla partecipazione. Il provvedimento pertanto non rimuove i vincoli di carattere strutturale, congeniti a tali forme societarie, così come non definisce un nuovo statuto normativo con un modello societario intermedio tra le società quotate azionarie e le società chiuse, capace di offrire maggiori Siamo quindi di fronte ad una riforma superficiale da questo punto di vista, che dimostra mancanza di visione e che rischia di vanificare l'obiettivo prefissato di facilitare la quotazione e la permanenza nel mercato finanziario delle PMI sotto forma di Srl. È come se in un gran premio volessimo far correre una Fiat 500 come una Ferrari, cambiando ruote e carrozzeria, ma lasciando inalterati i motori e l'assetto di marcia. Altro tema invece fondamentale del provvedimento in esame è il voto di lista del ossia la possibilità agli amministratori uscenti di presentare una propria lista in sede di rinnovo dell'organo amministrativo. Com'è noto, l'articolo 147-*ter* del TUF ammette il voto di lista, garantendo la rappresentanza dei soci di minoranza, ma non disciplina la possibilità per gli amministratori di proporre una propria lista. È una prassi, quella della lista del consiglio di amministrazione, richiamata dal codice di autodisciplina di *corporate governance* e tipica delle compagini societarie a capitale diffuso presenti anche in molti Paesi europei. Secondo Assonime in Italia sono 50 le società quotate, ovvero il 21 per cento, a prevedere nello statuto tale possibilità, ma sono solo 15 ad aver adottato tale scelta, tra cui Telecom Italia, Generali e UniCredit. Il tema, apparentemente solo tecnico, rischia di avere rilevanti effetti sul futuro del nostro capitalismo, perché finisce per mettere in discussione il primato degli azionisti di maggioranza relativa e tende a far accrescere la managerialità delle nostre imprese, favorendo così la loro progressiva apertura al mercato finanziario. La norma, nonostante la sua importanza e rilevanza, non risultava presente nel disegno di legge governativo, a dimostrazione ancora dell'approssimazione con cui il testo è stato redatto ed approvato dal Governo. Il MoVimento 5 Stelle, sin dall'inizio, si è posto a favore di tale opportunità, demandando agli statuti societari tale possibilità senza imporre schemi rigidi, viste le variegate situazioni di composizione societaria e soprattutto prevedendo tutele a favore della rappresentatività delle minoranze qualificate. Nonostante la sua introduzione, permangono criticità che potrebbero limitarne l'utilizzo e la diffusione, come la mancanza di definizione delle modalità di formazione della lista del CDA, la trasparenza dell'intero processo di composizione e la documentabilità delle decisioni. Non si prevedono inoltre strumenti per contenere il rischio dello strapotere dei *manager* uscenti che possono permanere senza fine all'interno della *governance* aziendale, limitando così il ricambio generazionale, che spesso è fonte di innovazione e crescita. Di fronte a queste criticità, abbiamo avanzato proposte purtroppo non accolte, come il limite al numero di mandati amministrativi cumulabili dai *manager* nella stessa società, così come contemporaneamente in altre società, nonché il limite al numero degli amministratori uscenti da inserire nella lista del CDA in modo da evitare liste fotocopie e favorire l'ingresso di nuovi e giovani *manager*. Sempre per limitare il possibile strapotere del del *management* abbiamo riproposto, anche qui senza esito, una disciplina che il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo per contenere gli stipendi stratosferici dei *top manager* *(Applausi)*, che in molte realtà, anche italiane, ha raggiunto cifre esorbitanti, superando persino di 600 volte quelli dell'ultimo lavoratore in grado. Lungi dal voler stabilire un tetto, che potrebbe essere fonte di fuga di cervelli, abbiamo proposto da tempo una norma ispirata al pensiero di Olivetti, che prevede il mantenimento di un rapporto cosiddetto di equità, fissato da uno a cinquanta tra lo stipendio del *top manager* e quello dei lavoratori di grado più basso. un provvedimento che contribuirebbe a far aumentare salari bassi, fermi da oltre vent'anni, migliorando allo stesso tempo la produttività. Per favorire la partecipazione qualificata dei lavoratori, abbiamo inoltre previsto la partecipazione al consiglio di amministrazione di un loro rappresentante di comprovata professionalità, esperienza e competenza nel settore. Ma anche questa proposta non è stata accolta dal Governo. tema di grande interesse, su cui la Commissione ha molto dibattuto, è stato il voto plurimo o multiplo, un vero dilemma, dove la maggioranza ha dimostrato tutte le sue divisioni. In particolare, per il voto plurimo a favore delle società non quotate il Governo ha preferito confermare la norma attuale, aumentando *sic et simpliciter* il voto da assegnare alle azioni a voto plurimo, innalzandolo fino a dieci voti. Tale scelta va in controtendenza rispetto all'obiettivo di rendere più aperto e attrattivo il mercato finanziario. finanziario. Per evitare abusi da parte dei soci di controllo e per rafforzare le tutele a favore di investitori istituzionali e risparmiatori, il MoVimento 5 Stelle ha preferito estendere anche alle società non quotate il sistema del voto maggiorato, con una premialità a favore dei soci stabili, per contrastare anche la speculazione. È uno strumento, quello del voto plurimo, poco democratico, che rafforza, senza condizioni di merito, solo l'azionista di riferimento, il quale continua a mantenere il controllo societario in maniera non proporzionale al capitale posseduto, con la conseguenza di limitare le tutele e gli interessi delle minoranze. Ancora una volta, Presidente, il Governo dimostra di essere vicino ai poteri economici, sacrificando però gli interessi del Paese e dei soci di minoranza. In questi termini si vanifica l'esigenza di rendere più attrattivo, aperto e competitivo il nostro mercato dei capitali. Infine, riguardo al sistema del voto maggioritario per le società quotate, la norma in esame prevede un'ulteriore maggiorazione rispetto ai due voti massimi previsti dall'attuale normativa. In questo caso noi abbiamo condiviso la prospettiva di aumentare il voto maggiorato, legandolo però al principio della stabilità dell'azionista. In ultimo, il provvedimento in esame prevede la delega al Governo per modificare il TUF. In definitiva, si vuole già riformare quello che oggi si approva: un'assurdità e un chiaro segnale dell'incapacità del Governo di racchiudere nel testo in esame le modifiche che ritiene necessarie per rilanciare il nostro sistema finanziario. Si rimanda così a un successivo provvedimento quello che oggi si ritiene già inutile. Le norme in approvazione, pertanto, rischiano di avere validità temporanea, di creare confusione e incertezza tra gli operatori e di destabilizzare il sistema finanziario per il carattere intrinsecamente transitorio delle norme. pur ritenendo validi gli intenti originari del provvedimento in esame, esprimo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione, non condividendo i risultati raggiunti nel loro complesso. Ancora una volta il Governo Meloni e la maggioranza dimostrano la loro incapacità e soprattutto la mancanza di coraggio nel riformare un settore strategico per la crescita del nostro Paese. è proprio con riferimento alla mancanza di coraggio, Presidente, che vorrei concludere questo mio intervento citando Seneca, che a riguardo di coraggio dice: «Non è perché le cose sono difficili

Signor Presidente, questo disegno di legge è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano infatti è ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate. Nel corso degli ultimi dieci anni mediamente solo quattro società all'anno sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale al PIL, si è attestata notevolmente Allo stesso tempo, nel 2018, il numero totale di obbligazioni societarie emesse in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane era stato pari a circa solo il 6 per cento di tutte le emissioni europee. Inoltre, il 90 per cento di tutte le obbligazioni societarie italiane era quotato in una borsa estera, mentre solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali italiani era investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane: un dato che evidenzia le dimensioni contenute del mercato italiano. Per contro, gli investitori italiani avevano allocato circa 190 miliardi di euro agli investimenti nel capitale di rischio di imprese oltreconfine. Infine, si pensi che i titoli italiani rappresentano circa il 3,6 di quelli europei, mentre i titoli francesi rappresentano circa il 18 per cento. Quindi, è evidente che il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali, sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di questa debolezza e ostacoli sono comuni all'intera area dell'Unione europea, che rispetto ad altre principali aree economiche a livello internazionale presenta un *gap* competitivo significativo, dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell'evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali. Il declino dei mercati azionari europei è stato accentuato rispetto a quello di altre principali piazze finanziarie: un *trend* che riguarda i dati del mercato sia primario che secondario. La dimensione del mercato azionario europeo è inferiore sia a quello nordamericano, sia a quello delle altre principali piazze finanziarie internazionali. Una parte delle debolezze denunciate con riferimento ai mercati di capitale è però specifica del contesto italiano e si riflette in uno spiazzamento competitivo del mercato dei capitali italiano anche rispetto ai mercati più dinamici dell'Unione europea. Quindi, prendendo spunto da questa che è una situazione generale, il provvedimento si è posto gli obiettivi di promuovere le nuove ammissioni alla quotazione e la permanenza sul mercato regolamentato soprattutto delle PMI; potenziare il ruolo degli organi di regolamentazione e consolidare il quadro istituzionale; migliorare le condizioni per la partecipazione da parte degli investitori individuali qualificati; incoraggiare la partecipazione ai mercati di capitali italiani da parte di investitori istituzionali; migliorare l'accesso alle condizioni di liquidità nel mercato delle obbligazioni societarie per le imprese non finanziarie; valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell'accesso al mercato e rendere il sistema di applicazione delle regole più efficace ed efficiente. Per far questo sono numerosissimi i provvedimenti che sono contenuti in questo disegno di legge. Cito i principali, che sono stati già oggetto di discussione e hanno catalizzato per molte settimane

che il numero dei candidati sia pari a quello necessario, maggiorato di un terzo, e che i posti in consiglio siano distribuiti in maniera proporzionale alle liste di minoranza che abbiano ottenuto più del 20 per cento, eliminando quindi il discusso super premio del 49 Un'altra importante innovazione è quella del voto maggiorato: le società potranno introdurre nei propri statuti, appunto, il voto maggiorato, arrivando fino a un moltiplicatore di dieci, dando quindi più potere agli azionisti stabili. I diritti di voto concessi agli azionisti cresceranno di anno in anno, con la possibilità di arrivare fino a un massimo di dieci voti per azione, che sarà quindi diluita nell'arco temporale di un decennio.

ben specifici: sostenere la crescita del Paese favorendo l'accesso delle imprese al capitale di rischio, con particolare riguardo ai mercati regolamentati; aumentare la competitività del mercato nazionale; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti; facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati; rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione; semplificare le regole del governo societario; prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni e assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative. Si tratta, quindi, di paletti e principi ben precisi che il Governo dovrà rispettare per riformare il TUF. Oltre a queste, che sono delle importantissime novità, ve ne sono molte altre. Ne cito alcune: ad esempio, il capo I introduce misure di semplificazione del quadro normativo e di incentivo al rafforzamento dei mercati di capitali. Ci sono degli interventi volti ad ampliare i casi di esenzione della disciplina dell'offerta fuori sede, ricomprendendovi anche l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi superiori o uguali a 250.000 euro e alle offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con il diritto di voto effettuate da emittenti quotate sui mercati regolamentati; viene innalzata da 500 milioni a un miliardo di euro la soglia di capitalizzazione rilevante ai fini della qualifica di piccola e media impresa; si consente alle piccole e medie imprese di accedere su base volontaria al regime di dematerializzazione previsto dal TUF, con emissione in forma scritturale delle quote. Viene riformata la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi che riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato di capitali. Trading Facilities, MTF) la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Viene prevista la soppressione della possibilità attribuita alla Consob di aumentare il flottante qualora un soggetto che detiene un'interessenza superiore al 90 per cento del capitale rappresentato dai titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento della quotazione. Con l'articolo 8 vengono riproposte alcune misure già introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020 per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitale italiane. In particolare, sono previsti, per un periodo sperimentale fino al 30 aprile 2025, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali. Viene introdotta poi una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione. Viene chiarito che i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della relativa bozza. Viene abrogato l'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo. Si consente, ove contemplato dallo Statuto, che le assemblee di società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. L'articolo 18 reca norme relative alla disciplina del *cooling* *off* o del *cooling in*, ossia regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato. Inoltre, l'articolo 21 mira a promuovere l'inclusione finanziaria nel nostro Paese inserendo l'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica. Purtroppo il tempo è troppo poco per citare tutte le

che ad oggi comunque è sottodimensionato e ha molti difetti. Ritengo che il lavoro che è stato fatto in Commissione dalla maggioranza, e in molti casi anche grazie all'aiuto dell'opposizione, abbia prodotto un testo che sicuramente porterà il mercato dei capitali italiano a essere al passo con quello dei maggiori

Signor Presidente, mi rivolgo per suo tramite soprattutto ai colleghi della maggioranza e ai membri del Governo - saluto il sottosegretario Freni - per rappresentare - come abbiamo già fatto in Commissione il nostro rammarico per il metodo, ancora prima che per il merito, con cui il Governo e la maggioranza parlamentare hanno condotto l'*iter* di questo disegno di legge e della delega collegata che - come abbiamo visto nella discussione - operano su materie di estrema delicatezza per la credibilità e l'affidabilità del Paese nel consesso economico e finanziario internazionale. Pensiamo che oggi avremmo potuto giungere a una convergenza di valutazioni più ampie sul testo che è approdato all'esame della 6a Commissione già la scorsa primavera.

con lo scopo evidente di semplificare e riformare la legislazione italiana, allineandola alle migliori prassi internazionali. Su quel testo si scelse di far esprimere, su impulso del MEF, della Consob, di Banca d'Italia, attraverso una consultazione pubblica, gli operatori di mercato e le associazioni di categoria, addivenendo infine alla pubblicazione nel 2022 del già citato Libro verde che, con ampio consenso degli operatori e degli osservatori del settore, si poneva alla base del processo legislativo; questo in maniera seria, trasparente e comprensibile dalle imprese e dagli investitori a livello internazionale. Noi riteniamo che quel percorso sia stato male interpretato dalla maggioranza che, talora mostrando imperizia e una certa estemporaneità, ha emendato il testo introducendo meccanismi macchinosi e farraginosi su temi delicati, quali sono quelli di cui abbiamo discusso (il voto di lista e la maggiorazione del voto), costringendo poi il Governo a numerose mediazioni e riformulazioni del testo. circostanza ha poi indotto osservatori e testate economiche a sospettare che la maggioranza si stesse muovendo non in difesa di un interesse generale, ma avendo a mente alcune situazioni particolari, cosa che mai deve succedere nel processo legislativo. *(Applausi)*. Grande perplessità suscita poi anche Grande perplessità suscita poi anche la quasi totalità di sovrapposizione della delega di riforma del testo unico della finanza (TUF) con il provvedimento che oggi votiamo. Basta leggere gli articoli della delega per capire che, contrariamente a quanto è stato sostenuto in quest'Aula, la sovrapposizione c'è anche sul tema della maggiorazione del voto. Ricordo a tutti noi che la certezza del diritto è precondizione essenziale per qualunque investimento che il disegno di legge capitali possa configurare una sorta di *temporary rule* - come si direbbe nel diritto anglosassone - cioè una legge a tempo destinata ad essere superata dalla delega, non è certo un buon viatico per rendere competitivo a livello internazionale il mercato dei nostri capitali. Nonostante queste considerazioni che - come avete ascoltato - sono fortemente critiche, nei lavori di Commissione non ci siamo mai sottratti dal proporre miglioramenti al testo, nello spirito costruttivo che ha caratterizzato il percorso della costruzione del Libro verde durante la scorsa legislatura. Risulta quindi inspiegabile come mai il nostro emendamento - l'ho illustrato in precedenza - che richiedeva la costituzione di un comitato tecnico composto da esperti di alto profilo internazionale per affiancare il Governo nell'attuazione della delega, sia stato respinto. Ricordo che lo stesso metodo fu adottato, nella sua veste di direttore generale del Tesoro, da Mario Draghi nel 1997 e nel 1998, quando il Testo unico sulle attività finanziarie tuttora vigente fu costruito. Furono un percorso e un esito che portarono al Paese credibilità e autorevolezza. Dobbiamo quindi pensare che il Governo abbia timore di avvalersi di esperti indipendenti su temi di carattere eminentemente tecnico? Voglio sperare sinceramente di no e, quindi, auspico ancora che, nel percorso che porterà questo provvedimento e la delega alla Camera e poi all'attuazione della delega da parte del Governo, si possa rimediare su questo La nostra volontà rimane collaborativa nell'interesse del Paese e della credibilità e stabilità economica dell'Italia, in un momento in cui tutti sappiamo che il Paese è un osservato speciale sui mercati internazionali per via dell'importante e crescente debito pubblico. Anche misure di questa natura, che possono sembrare tecniche, vengono osservate con un occhio particolare da investitori e imprese a livello internazionale. Quelle appena illustrate sono le ragioni per cui, pur confermando uno spirito collaborativo

i provvedimenti in discussione e che andremo ad approvare portano seco due importanti segnali di discontinuità con il passato: il diritto alla conoscenza delle regole della finanza e la necessità di adeguare il contesto normativo del Paese alle regole europee, tenendo però in considerazione la realtà economica del Paese; il suo tessuto imprenditoriale, fatto di piccole e medie imprese e il loro valore umano prima ancora che economico; le famiglie che tante volte sono dietro a tali imprese. Sono argomenti molto cari alla nostra parte politica. un cambio culturale, dunque, frutto di una mentalità liberale che è difficile rinvenire se non andando in là con gli anni. se ripercorriamo i sessant'anni che ci separano dalla svolta del 1962, è difficile non stupirsi di fronte all'incredibile continuità delle scelte delle nostre classi dirigenti in materia di istruzione, quale che ne fosse il colore politico. È altrettanto paradossale che le innumerevoli riforme che hanno investito la scuola declinassero spaventosamente verso una rimozione delle barriere del merito e una facilitazione esasperante degli studi, quasi a valorizzare la non conoscenza, ovvero il trionfo dell'anarchia. È chiaro che dentro questa cornice generale veniva a sfumare, fino poi a sparire e ad annullarsi, l'insegnamento dell'educazione civica, perché non vi è la cultura di far crescere lo studente come cittadino di domani Peggio ancora: vi era la volontà di mantenere l'ignoranza su taluni argomenti che, anche nell'immaginario collettivo, erano destinati a pochi per scelta politica. La finanza è l'archetipo di questa *forma mentis*, diretta a consegnare a pochi eletti le regole del gioco, per escludere scientificamente la collettività. Oggi il Parlamento istituisce l'educazione finanziaria come materia di studio, affinché sin dagli albori del percorso formativo si consenta alle nuove generazioni di essere informate sugli strumenti che concorrono allo sviluppo del Paese l'abitudine a conoscere per decidere, che è la base per ogni società che si definisca, nei fatti e non nelle parole dei simboli dei partiti, democratica. Questo non significa omologare e massificare la conoscenza, tutt'altro. L'ambizione dichiarata è quella di dare la possibilità a tutti di essere sui blocchi di partenza e non limitare a pochi la possibilità di correre i cento metri. Sarebbe riduttivo e a tratti ingenuo limitarsi però a enfatizzare solo la portata, anche se storica, dell'articolo 21. Questa proposta di legge, infatti - come ho detto nelle premesse - costituisce il culmine di un processo di consultazione cominciato con il *report* "Capital Market Review of Italy" dell'OCSE, sviluppatosi nel Libro verde del 2022. La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita non può essere effettiva se anche questo importante settore non si armonizza con gli altri interventi, primi fra tutti quelli dei fondi del PNRR. Cito la rimozione dei vincoli, sia legali che operativi, all'accesso al mercato delle imprese, incentivando nella loro direzione il risparmio dei privati, con un effettivo controllo: semplificare è giusto e doveroso, ma è altrettanto doveroso approntare degli strumenti per evitare - come è capitato in passato - che alla semplificazione corrispondesse quel "libera tutti" che abbiamo letto nei giornali e visto nei tribunali. Oltre a ciò, segnalo l'importantissima riforma organica della disciplina delle società emittenti di strumenti finanziari diffusi, la soppressione di molteplici obblighi che accomunano tale categoria di società a quelle con titoli quotati in mercati regolamentati. L'eliminazione di questi obblighi garantisce maggior facilità di circolazione del loro capitale, mantenendo comunque adeguato il livello di garanzia degli operatori. L'obiettivo ultimo, in sostanza, è costituire un gradino normativo che permetta al sistema finanziario di diversificarsi in relazione alle diverse esigenze di tutela degli investitori e società differenti. Infine, ma non per questo destinati a essere solo un titolo di coda, vi sono gli interventi significativi in materia di piccola e media impresa. La proposta di legge riporta queste società al loro giusto alveo, quello del motore di un Paese dove le PMI costituiscono l'ossatura del tessuto economico, al quale attribuire la giusta dignità e non solo un ruolo troppo spesso ancillare. Questa dignità passa, anche e soprattutto, nell'innalzare la capitalizzazione massima delle PMI a un miliardo di euro e nel semplificare l'ammissione alla quotazione. Come anche si registra l'importanza non banale della possibilità di conferimento delle deleghe di voto ai gestori di portafogli. L'eliminazione del riferimento al conferimento di tali deleghe per singole assemblee implica la possibilità di rilasciarle per molteplici occasioni. In tal modo, oltre a favorire l'esercizio dei diritti di *voice* degli azionisti, fondamentali per le società sane, viene riallineata la disciplina italiana al nuovo quadro normativo euro-unionale. È altresì degna di nota la riforma dell'articolo 2351 del codice civile, volta a delineare la flessibilità della disciplina italiana agli *standard* europei. La proposta, infatti, prevede l'incremento da tre a dieci del numero di voti assegnabili alla singola azione a voto plurimo e a partire dalle nuove quotazioni. Corredano la proposta numerose disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativo finanziari, limite alle emissioni di titoli di debito in materia di potere, anche sanzionatorio, della Consob e di tutela contro le frodi. Consentitemi poi lo sfogo, caratteristica che mi contraddistingue: troppo spesso si è alzato un coro stonato, nel *mainstream*, di coloro che, non avendo argomenti propri, ripetevano come un disco rotto l'incapacità di Fratelli d'Italia di rispettare le regole del Trattato dell'Unione. Ci trattavano da irresponsabili,

anche e soprattutto valutando le realtà economiche dello Stato, la spina dorsale del sistema Italia. Ed è questo il senso concreto della proposta di legge su cui, convintamente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore. Agli altri lasciamo il diritto di ragionare sulla lunghezza delle orate, sulle dimensioni delle melanzane, sul potere alimentare delle cavallette: a ciascuno il suo. Colleghi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16-*ter*.200,

la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico

Due giorni fa era l'anniversario - il quattordicesimo - della sua uccisione, per la quale - come è noto - ci sono state sentenze definitive che hanno dimostrato come lo Stato democratico può e deve essere capace di punire anche chi tra coloro che dovrebbero essere i suoi servitori viola leggi, norme, diritti umani e principi costituzionali. Del resto, chiedere scusa e colpire responsabili di violazioni è per uno Stato segno di forza e non di debolezza. La sorella Ilaria si è battuta per anni per la verità e la giustizia sull'uccisione di Stefano, un ragazzo che non doveva morire ucciso a trentuno anni mentre era sotto la custodia dello Stato. E lo ha fatto contro false testimonianze, omertà, comportamenti che sono stati sconfitti dal suo dolore; un dolore trasformato in coraggio, come quello dei suoi genitori, del suo avvocato Anselmo e quello di tante persone e associazioni, forze ed esponenti politici che l'hanno accompagnata in questa battaglia. E faccio un nome su tutti, quello di Luigi Manconi. preso però la parola, Presidente, anche per altre due ragioni che espongo brevemente. La prima è per esprimere solidarietà a Ilaria Cucchi *(Applausi)*, fatta oggetto di nuove minacce che lei ha denunciato proprio in questi giorni. Le siamo vicini contro l'odio e gli *stalker*. poi ringraziarla. Sì, la voglio ringraziare per l'onore e la disciplina con i quali svolge il suo mandato parlamentare. La battaglia nel nome di suo fratello Ilaria la conduce ancora, tutti i giorni; ne siamo testimoni in Commissione giustizia, lo vediamo con il suo recarsi a visitare carceri e verificare le condizioni dei detenuti. A questo proposito, Presidente, unisca anche lei la voce, assieme alla nostra e a quella di tutti, per la vera e drammatica emergenza carceri. Lo abbiamo visto altresì con il suo recarsi a visitare per esempio, nei giorni scorsi, il di Ponte Galeria, a ispezionare quella struttura dove degli esseri umani, scappati da fame, miseria, persecuzioni, guerre e mancanza di futuro sono reclusi e trattati come gli esseri umani non dovrebbero mai essere.

avere certezze. Ho finito. Ho voluto dire queste cose per ricordare innanzitutto la morte di Stefano Cucchi, ma anche per ringraziare la senatrice Cucchi che fa vivere il ricordo di suo fratello ogni giorno, anche con intransigente passione, attraverso valori e principi che tutti noi dovremmo condividere e provare a far vivere.

che forse in questo Parlamento dovremmo discutere di più per capire come affrontare e dare risposta a problemi che abbiamo tutti noi come società. Grazie Ilaria.

che certo la senatrice Ilaria Cucchi sta facendo insieme a noi, ma che io credo debba essere considerato un patrimonio del Senato intero. L'idea che, quando un nostro concittadino è nelle mani delle autorità,

ha dato sostanza alla personalità dei cittadini e ha messo fine all'arbitrio del potere. Io credo che la storia di Stefano Cucchi esemplifichi che cosa tutto questo significa, che cosa significa vivere in uno Stato democratico, essere in custodia di quello Stato e avere la garanzia che lo Stato saprà irrogare sanzioni penali se quel quel cittadino ha commesso reati; ma in ogni caso quelle sanzioni penali non saranno mai rivolte contro la dignità umana di quella persona. Uno Stato democratico è questo: lo Stato nel quale i cittadini delegano l'uso della forza e della coercizione allo Stato e lo Stato risponde a quella delega nel sacro impegno di esercitarla entro i limiti della legge e della Costituzione. La storia di Stefano Cucchi ci racconta che non sempre è così, che purtroppo ancora oggi in molti casi sentiamo parlare di maltrattamenti. Sono aperte procedure penali nei confronti di persone che dovrebbero rappresentare lo Stato. E io credo che, proprio nell'interesse di chi invece serve lo Stato con fedeltà ai principi della Costituzione, non dobbiamo dare nessun margine di operatività, nessun margine di libertà a chi vìola quei principi che - ripeto - a mio avviso hanno il carattere della sacralità. Utilizziamo questi momenti e questa data certo per ricordare Stefano, certo per ringraziare Ilaria - permettimi di chiamarti così - ma soprattutto per ricordare che la sua battaglia, la loro battaglia, ha una valenza universale che va ben al di là del caso specifico. Signor Presidente, ci è parso doveroso e necessario cogliere l'occasione, per me preziosa, di ringraziare Ilaria Cucchi. Lo faccio a titolo personale e a nome del Gruppo politico che rappresento, nel ricordo naturalmente del fratello Stefano Cucchi. Ricordo vividamente quella vicenda, che il nostro Paese ha attraversato e ha segnato davvero alcune delle pagine più cupe, anche dal punto di vista di alcune comunicazioni e dichiarazioni istituzionali che sono state rilasciate in quel periodo. Ma andiamo avanti, non rivanghiamo quel passato. Io sento di dover ringraziare Ilaria Cucchi, perché ha evitato un pericolo a questo Paese. Se non fosse stato per la sua la sua determinazione, per la sua forza e per il suo coraggio incrollabile nella ricerca della giustizia e nella ricerca semplicemente di rimettere le cose al proprio posto, posto, individuando le responsabilità là dove ce ne sono, al di là di chi siano e che ruoli ricoprano i responsabili, io credo che il nostro Paese ne avrebbe riportato un danno enorme. Invece, grazie all'impegno di Ilaria e di chi le è stato accanto, questo pericolo il nostro Paese lo ha scampato. Oggi possiamo dirci più orgogliosamente dalla parte delle istituzioni e dalla parte delle Forze dell'ordine, che certamente hanno guadagnato da questa azione di pulizia, trasparenza e identificazione delle responsabilità. Come è stato già detto in precedenza, chiunque è nelle mani dello Stato deve essere doppiamente garantito e doppiamente protetto, e non il contrario. Mi unisco, quindi, ai ringraziamenti di chi ha parlato prima di me nel ricordo di Stefano Cucchi.